concittadino, Mario Carmine Paciolla, è stato trovato privo di vita in Colombia, Paese dove si trovava per conto delle Nazioni Nell'esprimere le nostre condoglianze alla famiglia, chiediamo al Governo di intraprendere tutte le iniziative necessarie perché si faccia luce, per conoscere la verità di questo ragazzo. Le chiedo, signor Ministro, di pretendere - sì, è questa la parola giusta - dalle Nazioni Unite la massima collaborazione con le autorità italiane e con i legali della famiglia di Mario Carmine Paciolla. Da quanto mi risulta, infatti, c'è da parte dei responsabili dell'ONU un silenzio assordante. Il 15 luglio, una settimana fa, Mario Carmine Paciolla, napoletano di trentatré anni, viene trovato privo di vita presso la propria abitazione a San Vicente del Caguán, località a 650 chilometri da Bogotà. Il connazionale era un cooperante ONU ed era impegnato da due anni con le Nazioni Unite in un progetto che mirava a riconvertire gli ex combattenti al lavoro nei campi e svolgeva il monitoraggio per il rispetto degli accordi di pace tra il Governo colombiano e le FARC (forze armate rivoluzionarie della Colombia). Da quanto si apprende dalla stampa locale, le autorità colombiane all'inizio hanno parlato di suicidio, circostanza che non ha trovato riscontro, smentita dalle testimonianze delle organizzazioni cooperanti in Colombia e dalla stessa famiglia del giovane. Sul cadavere di Mario Carmine Paciolla, come riportano gli organi e le agenzie di stampa, ci sarebbero evidenti segni di violenza, in particolare tagli provocati da coltelli o da lame acuminate, che non sono state trovate in casa. Sappiamo che in Colombia è stata effettuata l'autopsia, alla quale ci risulta abbia partecipato un medico indicato dalle Nazioni Unite. All'autopsia non ha però potuto partecipare il perito di parte della famiglia Paciolla. L'11 luglio, nel corso di una telefonata intercorsa tra Mario - il ragazzo napoletano - e la madre, egli aveva manifestato una certa preoccupazione per alcune cose accadute, un «qualcosa di strano», per «un guaio» non meglio specificato, e il 20 luglio sarebbe voluto tornare in Italia. Signor Ministro, Napoli è mobilitata per conoscere la verità su questa storia: pensi soltanto che sui balconi del municipio c'è uno striscione e che sulla

Signor Presidente, senatrici e senatori, il connazionale Carmine Mario Paciolla, come ricorda il senatore Ruotolo, è stato trovato senza vita lo scorso 15 luglio nella sua abitazione a San Vincenzo del Lì lavorava dal 20 agosto 2018 come volontario ONU nella missione di verifica chiamata a monitorare l'attuazione dell'accordo di pace del 2016 tra il Governo e le FARC, i guerriglieri delle forze armate rivoluzionarie della Colombia. abbiamo seguito con la massima attenzione questa dolorosa vicenda. La nostra ambasciata a Bogotà mantiene un costante contatto con le autorità colombiane e con i familiari del connazionale, ai quali sta prestando ogni possibile assistenza, e la Farnesina ovviamente incoraggia l'ONU a fare il massimo anche in tal senso. Le indagini della polizia locale per chiarire le cause della morte sono in corso. Le autorità colombiane ci hanno assicurato che il caso, di cui subito abbiamo sottolineato il massimo rilievo, è anche da loro ritenuto di assoluta priorità ed è seguito al più alto livello direttamente dal procuratore generale della Nazione e dalla sua vice. I colombiani hanno inoltre nominato un magistrato specializzato per curare queste indagini con l'impiego di investigatori esperti e di un *team* speciale forense inviato sul posto da Bogotà per giungere nel più breve tempo possibile alla verità su quanto accaduto. È stata effettuata l'autopsia il 17 luglio e ne attendiamo nei prossimi giorni i risultati. L'ambasciata si è attivata per espletare tutte le pratiche necessarie per il rimpatrio della salma del giovane connazionale, che arriverà domani qui in Italia. Assicuro il massimo impegno della Farnesina e mio personale nel seguire questa tragica vicenda, che ha coinvolto un nostro giovane brillante, impegnato in una missione molto delicata. La sua prematura scomparsa suscita giustamente l'attenzione dell'opinione pubblica e di questo Parlamento. Vorrei dire che siamo vicini ai suoi familiari in questo triste momento e non risparmieremo alcuno sforzo finché non verrà fatta piena luce su quanto gli è accaduto.

se si fosse suicidato, che senso avrebbe avuto chiamare la madre, che non sentiva spesso, e prepararsi il viaggio di ritorno? Ecco perché dobbiamo fugare qualsiasi dubbio

Ministro, per la celerità con cui è venuto a riferire qui in Senato su questa triste vicenda. Solo martedì in quest'Aula avevo chiesto un suo intervento per informare il Parlamento, annunciando questa interrogazione. La sua presenza oggi testimonia l'attenzione e la sensibilità del suo Ministero verso i nostri cittadini italiani all'estero. Purtroppo questa storia triste ha davvero diversi tratti di ambiguità. Mi permetto di ricordare che Paciolla era inquadrato nella missione ONU per il monitoraggio dell'accordo di pace tra FARC e Governo colombiano e il nostro cooperante si trovava in un'area particolarmente pericolosa del Paese. Pochi giorni prima della sua morte aveva manifestato a familiari e amici timori per la sua vita, tanto da aver acquistato sollecitamente un biglietto aereo per il 20 luglio: l'intento di Mario era quello di tornare a casa. Risulta perciò opinabile che un cooperante con esperienza decida di suicidarsi proprio qualche giorno prima di rientrare in Italia e per di più senza un apparente motivo. A quanto pare, secondo quanto riportato da alcuni *media* locali, sul corpo di Mario sono state riscontrate ferite da taglio. Ovviamente è necessario attendere i risultati ufficiali dell'autopsia per conoscere con certezza il reale motivo del decesso, ma ripeto che temo ci siano ancora delle ombre su cui far luce. Signor Ministro, dalla firma dell'accordo di pace tra FARC e Governo colombiano ad oggi sono quasi mille i morti assassinati: attivisti per i diritti umani, indigeni, contadini ed ex miliziani delle FARC che erano stati reinseriti nel tessuto sociale colombiano, una vera e propria strage su cui la comunità internazionale, di solito molto attenta ai diritti umani nell'area, non ha speso una parola. Queste ragioni, signor Ministro, mi portano a porle alcune domande più precise: a che punto sono le indagini? Si riscontra una piena collaborazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle autorità colombiane? Quali attività sono state intraprese per facilitare il rientro della salma in Italia e quali iniziative ha adottato per promuovere la più proficua collaborazione tra l'autorità giudiziaria italiana e quella colombiana? *(Applausi)*.

il Parlamento intenda sottolineare l'importanza e l'urgenza di chiarire le circostanze della tragica fine del giovane volontario le Nazioni Unite Carmine Mario Paciolla e questo è naturalmente anche l'obiettivo del Governo. Abbiamo attribuito priorità a questa triste vicenda, che seguo personalmente venendo costantemente aggiornato sui suoi sviluppi. La nostra ambasciata a Bogotà è in contatto sia con la famiglia Paciolla, cui sta prestando la massima assistenza, sia con le autorità colombiane e con gli inquirenti, sotto la guida del procuratore generale di quel Paese. Le indagini si svolgono con l'ausilio di un magistrato specializzato in questo tipo di delitti e di una squadra di tecnici forensi. Le cause del decesso sono ancora poco chiare. Siamo in attesa dei risultati delle due autopsie, sia quella effettuata dall'autorità colombiana sia quella che verrà eseguita su disposizione dell'autorità giudiziaria italiana. Ovviamente saranno cruciali anche tutte le testimonianze. La missione delle Nazioni Unite in cui Carmine Mario lavorava ha l'obiettivo di verificare il reinserimento degli ex guerriglieri delle FARC nella vita politica, economica e sociale della Colombia, nonché le garanzie di integrazione, sicurezza e protezione per le loro famiglie e le comunità coinvolte. La nostra rappresentanza presso le Nazioni Unite a New York ha effettuato un passo con il responsabile del dipartimento competente per la missione di verifica ONU in Colombia. Abbiamo sottolineato la ferma aspettativa di una continua e piena collaborazione da parte della missione con la nostra ambasciata a Bogotà e ci è stato confermato che è stata avviata un'indagine interna, che vede per il momento impiegate capacità investigative della stessa missione ONU. Abbiamo chiesto e ottenuto che sia condotta in maniera rapida e approfondita. Gli esiti saranno tempestivamente condivisi con la nostra ambasciata a Bogotà e con la rappresentanza a New York. Quindi, per ricapitolare, saranno fondamentali tre linee di inchiesta: quella colombiana, quella delle Nazioni Unite e quella della magistratura italiana. Il lavoro della Farnesina sarà quello di garantire il massimo coordinamento tra le attività delle autorità coinvolte e su questo vi assicuro la massima tempestività e il massimo impegno. Vi informo, peraltro, che intendo incontrare quanto prima la famiglia Paciolla per esprimere personalmente la vicinanza dello Stato italiano; vicinanza che continuerà senza interruzione, anche lontano dai riflettori, fino a che non verranno chiariti tutti i contorni della morte di Carmine Mario Paciolla, nostro concittadino. ministro Di Maio, la ringrazio per la sua risposta. Credo che lei oggi qui stia dimostrando una lodevole premura per questo triste caso. Auspico che i parenti e gli amici di Mario, seppur nel dolore, essere rassicurati dalla vicinanza delle istituzioni che lei e noi tutti rappresentiamo. In questo tempo complesso la politica estera italiana, forse come poche volte nella storia repubblicana, sta dimostrando grande attenzione verso i tanti italiani presenti in ogni continente. Penso alla determinazione e all'efficienza che lei ha dimostrato durante l'emergenza Covid sia impegnandosi a reperire l'indispensabile materiale sanitario sia assistendo i tanti connazionali bloccati in molti Paesi. Senza l'incessante lavoro degli uomini e delle donne della Farnesina, migliaia e migliaia di connazionali non sarebbero potuti tornare in Patria. Concludo, signor Ministro, ricordando che se il nostro Paese è tanto ammirato e considerato è anche per il lavoro dei nostri cooperanti, che operano con coraggio nei campi profughi accanto a chi soffre, nell'interposizione in aree di conflitto, nella ricerca costante del dialogo e della pace, anche a costo della propria vita. A loro vanno tutto il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine, consapevoli che, se l'Italia è un Paese particolarmente amato, è anche in virtù dei loro alti ideali di giustizia di cui siamo particolarmente orgogliosi.

signor Ministro per essere presente perché l'interrogazione che, come Fratelli d'Italia, abbiamo scelto oggi di presentare è drammatica. Un'intera Regione, la Liguria, è veramente isolata ed è diventata un'isola: non c'è più la possibilità di una circolazione stradale che abbia anche solo lontanamente il requisito della normalità. Da due anni, come tutti sanno, è crollato il ponte Morandi; dopo quello c'è stata una problematica e devo dire che l'assessore Balleari e la Giunta di Genova vi avevano in parte rimediato, con una strada fatta in soli due mesi. Adesso però la situazione delle autostrade è diventata drammatica: c'è un'interruzione continua, si viaggia a una sola corsia con code chilometriche e tempi di percorrenza impossibili. impossibili. Come se ciò non bastasse, si è pure aggravata la situazione perché non vengono fatti i lavori sull'unica sull'unica strada alternativa, la via Aurelia, dove piccole frane non vengono riparate da mesi e altri lentissimi lavori in corso rimangono a bloccare o a rendere assai difficoltosa anche la circolazione. tale situazione, se non la principale, è che essendo stato avviato da parte della società autostrade, con tutti i difetti che comporta,

reale e immediato abbiate in mente per salvare, nella stagione turistica in particolare, la Liguria e tutto il Nord Ovest da questa drammatica situazione.

Grazie dello stato di funzionalità delle infrastrutture, da effettuarsi secondo le modalità di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6736 del 19 luglio 1967, pienamente efficace e vincolante per tutti i concessionari. In particolare, il concessionario deve ispezionare, durante la sua normale attività quotidiana, i manufatti e le opere d'arte, mediante un esame di superficie delle strutture visibili (pile, pilastri, colonne, archi, eccetera), tendente ad accertare ogni fatto nuovo e l'insorgere di eventuali anomalie esterne. Detta ispezione deve essere effettuata, in ogni caso, con scadenza almeno trimestrale e mediante l'elaborazione di un *report* recante i principali dati e le risultanze delle verifiche. Inoltre, il concessionario deve effettuare, con cadenza annuale, un esame generale e completo dei manufatti più importanti, anche mediante saggi ed ispezioni. Per quanto riguarda il sistema viario ligure, basato soprattutto sulla rete autostradale, nello scorso mese di gennaio la società Aspi ha presentato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma di ispezioni delle gallerie esistenti lungo tutta la tratta da essa gestita da attuare nel corso dell'anno 2020. È stato immediatamente segnalato e più volte ribadito in forma scritta alla società Aspi che il contenuto del programma ispettivo presentato doveva ritenersi integrativo e non già sostitutivo delle attività che la stessa era tenuta ad espletare in forza della circolare del 1967 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali. Conseguentemente la società Aspi ha proceduto a una riprogrammazione delle attività, prevedendo anche lo smontaggio degli elementi contenuti nelle gallerie, le cosiddette onduline. Tale attività ha determinato la chiusura temporanea di gallerie per l'effettuazione degli interventi di riparazione. Al fine di ridurre i disagi per l'utenza derivanti dall'attività ispettiva, il Ministero ha immediatamente avviato costanti interlocuzioni per individuare, anche d'intesa con la Regione Liguria e enti locali, che hanno sempre partecipato e presenziato ai tavoli tecnici, le modalità per l'espletamento della stessa. Con circolare del 7 luglio si è inoltre provveduto ad impartire indicazioni aggiornate sulle ispezioni ed è stata prevista la possibilità ulteriore di attivare, da parte dell'autorità prefettizia, un apposito tavolo di coordinamento per il monitoraggio dei fattori critici derivanti dall'effettuazione delle ispezioni e per l'individuazione di tutte le misure occorrenti per il loro superamento. Entro il prossimo 28 luglio saranno completate le verifiche e gli interventi e ripristinate le normali condizioni di viabilità. Confermo, senatore La Russa, che si sono verificati disagi molto gravi per l'utenza e lunghe attese per effettuare gli spostamenti sulla rete autostradale ligure. non possa essere messa in discussione, anche dopo i recenti fatti, la convinzione che la sicurezza delle infrastrutture, considerate le gravi condizioni delle gallerie in Liguria, costituisca un presupposto imprescindibile per garantire l'effettività del diritto costituzionale alla mobilità.

sicuramente il diritto alla sicurezza viene avanti a tutto, ma forse sarebbe stato bene che il Ministero non aspettasse otto mesi per intimare, il 20 maggio, che i lavori che si stavano svolgendo dall'inverno del 2019 erano, secondo il Ministero, diversi da quelli prescritti. Forse toccherà alla procura di Genova, presso cui è stato aperto un fascicolo a seguito dell'esposto del presidente della Regione Toti, verificare quali siano state le inadempienze della società Autostrade e del Governo. Quello che è sicuro è che lei mi ha dato una serie di risposte che giustificano l'attuale situazione, dicendo che ci sono verifiche, incontri ed interlocuzioni, ma non mi ha dato nessuna speranza che questo fine settimana o il prossimo la situazione cambi. La Liguria è veramente stretta in una morsa di intralci autostradali e stradali. Non mi ha parlato poi della situazione dell'Aurelia, anch'essa semi-impraticabile, che provoca un danno non solo alla Liguria e alla stagione turistica. Ma lei sa che il porto di Genova serve tutta la parte Nord dell'Italia? È un danno incalcolabile in cui il palleggiamento di responsabilità tra la società Autostrade e il Ministero ci lascia sconcertati, come sconcertante è l'assenza di una prospettiva seria di rimediare a questo disastro che avete combinato.

per essere qui. Tra le conseguenze negative derivanti dalla drammatica pandemia da Covid-19 emerge in maniera preponderante la riduzione dei consumi e anche la minore propensione, ovviamente, da parte dei cittadini ad andare in vacanza. Questo per la contrazione dei redditi, per le difficoltà economiche oggettive del Paese e anche, ovviamente, per le restrizioni che hanno riguardato soprattutto i rapporti con le altre Nazioni e, quindi, per quanto riguarda i viaggi intercontinentali, le restrizioni che hanno determinato lo stop ai viaggi in questo periodo. Secondo studi e dati forniti dal Codacons, un italiano su due si ritaglierà degli spazi per le vacanze. Questi spazi saranno orientati prevalentemente a viaggi all'interno del nostro Paese; viene stimato, appunto, che la gran parte dei cittadini che si muoveranno lo farà all'interno del Paese. Tra l'altro come stato anche manifestato da alcune associazioni, tra cui e altre società, come Bain & Company, la maggior parte degli spostamenti avverrà attraverso l'utilizzo dell'automobile e, molto spesso, anche attraverso il noleggio. Consideriamo quindi importante questo tema. È sicuro che la possibilità della ripresa degli spostamenti sarà un evento che dobbiamo accompagnare. Occorre considerare che, per quanto riguarda il sistema dei pedaggi autostradali, lo scorso anno l'Autorità di regolazione dei trasporti aveva emanato delle delibere relativamente all'adozione di un modello nuovo di fissazione delle tariffe, attraverso il metodo *price cap* (metodo che dovrebbe collegare la definizione della tariffa alla qualità del servizio in maniera più stretta).

descritte in premessa e se non ritenga opportuno adottare nel più breve tempo possibile tutte le iniziative di sua competenza volte a ridurre le tariffe autostradali, al fine di favorire i cittadini per quanto riguarda la mobilità,

trasporti*. Signor Presidente, gli atti convenzionali delle concessioni autostradali prevedono un aggiornamento quinquennale dei piani economico-finanziari, cosiddetti PEF. In occasione di ciascuna aggiornamento si provvede all'adeguamento del piano degli investimenti, alla riprogrammazione dei parametri tecnici, nonché alla

concessioni autostradali. Inoltre, in osservanza al nuovo contesto di riferimento, è stato chiesto alle società concessionarie di predisporre PEF conformi alla nuova disciplina tariffaria. Il decreto legge n. 162 del 2019 ha previsto una dettagliata tempistica per la presentazione di proposte di PEF da parte delle concessionarie autostradali, stabilendo anche il perfezionamento dell'*iter* approvativo entro il 31 luglio 2020. Come è noto, le misure di contenimento Covid-19 hanno determinato, però, un allungamento dei tempi previsti per la valutazione dei piani economico-finanziari. Il medesimo decreto-legge ha congelato gli incrementi tariffari per la quasi totalità della rete autostradale relativi all'anno 2020, e fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei PEF. Ad oggi, dunque, per l'anno 2020 non vi è stato e non vi sarà alcun incremento tariffario. Concludo evidenziando che, nella valutazione dei piani economico-finanziari, si terrà conto dell'equilibrio economico-finanziario e delle esigenze di favorire la mobilità sul territorio nazionale, in particolare laddove dovessero esserci aperture di cantieri che possono rallentare l'incedere del traffico, anche utilizzando politiche tariffarie coerenti con gli effetti economici determinati da Covid-19.

È un dato positivo il fatto che non ci saranno incrementi per tutto il 2020: è una buona notizia - anche se conosciuta - per i cittadini, che quindi non rischieranno un aggravamento dei costi per quanto riguarda la circolazione. È importante altresì in questa fase - sicuramente il Ministro lo farà,

le politiche tariffarie alla qualità dei servizi, secondo il principio chiave del *price cap.* Seguiremo la vicenda con attenzione sempre nell'ottica - comune a

al contempo di impiegare capitali comunque pubblici. Cassa depositi e prestiti ha una funzione particolare; il debito di Cassa depositi e prestiti è debito pubblico a tutti gli effetti, e non risulta che in Cassa depositi e prestiti ci siano le professionalità necessarie per gestire una macchina complessa come Autostrade per l'Italia, che è una delle più importanti aziende italiane dal punto di vista sia

svolgono la loro attività. Pertanto, è il sistema Italia nel suo insieme che viene danneggiato nel caso in cui la situazione non sia conveniente. E la situazione migliore conveniente ci sarebbe con una competizione.

nei confronti di Aspi, ricordo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 luglio scorso, ha esaminato le due proposte transattive trasmesse da parte di Aspi e Atlantia e ha ritenuto di avviare l'*iter* previsto dalla legge per la formale definizione di una transazione. Inizio dall'ultima richiesta fatta. La decisione di avviare la transazione - e non la procedura di revoca - ha determinato la continuità del rapporto concessorio tra lo Stato - il concedente (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) - e Autostrade per l'Italia. Nel caso si fosse addivenuti a una revoca,

per poi avviare, sui quattro lotti minimi previsti dalle nuove normative, lo svolgimento di autonome procedure di gara, i cui tempi previsti - considerato che c'è solo un precedente di conclusione nel nostro Paese - sono valutabili in tre o quattro anni. In questo tempo intercorrente per l'assegnazione della concessione non si sarebbe potuta ovviamente svolgere una serie di attività, tra cui rientrano le manutenzioni, gli interventi per la sicurezza e anche gli investimenti. Quindi, il rapporto concessorio è in continuità, mentre si modificheranno, alla luce delle proposte pervenute al Consiglio dei Ministri, gli assetti societari di Aspi. La soluzione individuata dal Consiglio dei ministri garantisce la piena realizzazione

(anche per le questioni di sicurezza) e la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo - nel contempo - una mole imponente (pari a 14,5 miliardi di euro) di nuovi investimenti. Preciso, alla luce della seconda domanda fatta, senatore Malan, che l'ingresso di Cassa depositi e prestiti non determina una statalizzazione di Aspi, dal momento che si prevede l'ingresso di nuovi investitori privati, ma consentirà di velocizzare il processo di trasformazione della società in una *public in una *public company* e il reperimento, pertanto, sul mercato, di ulteriori risorse per potenziare le infrastrutture e rafforzare anche il piano degli investimenti.

deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e, dunque, di procedure quantomeno pubbliche, mentre il gradimento di Cassa depositi e prestiti davvero ci rassicura poco. In ogni caso sarà necessario

In particolare, si chiede di conoscere i dettagli della proposta, con riguardo soprattutto alle quote di capitale che saranno acquistate da Cassa depositi e prestiti e da altri eventuali investitori. degli eventuali investitori - se si sa qualcosa, se ci sono dei paletti - e di sapere chi tra Cassa depositi e prestiti e gli altri eventuali investitori, ivi compresi quelli che sono già detentori di quote di Autostrade per l'Italia, avrà poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa

prestate in ordine all'effettiva realizzazione della manutenzione e degli investimenti previsti e all'effettiva riduzione dei pedaggi, specialmente in termini di compatibilità con la redditività dell'operazione per Cassa depositi e prestiti; se gli investimenti compensativi per 3,4 miliardi di euro previsti dalla proposta transattiva saranno realizzati prima o dopo l'ingresso di Cassa depositi e prestiti nel capitale di Autostrade per l'Italia SpA i dettagli del futuro piano industriale della "nuova" Autostrade per l'Italia SpA, anche rispetto ad un una futura revisione del sistema delle concessioni autostradali.

dagli altri colleghi senatori in questa seduta, sono a confermare che, per quel che riguarda l'assetto societario di Autostrade per l'Italia, l'azionista Atlantia si è reso disponibile, con formale lettera trasmessa ai Ministeri competenti, all'aumento di capitale da parte di Cassa depositi e prestiti. Questo implica che non ci sarà alcun passaggio di denaro tra

quotazione in borsa e, quindi, con la possibilità degli italiani e delle italiane di acquistare le azioni di Autostrade per l'Italia. Per quanto riguarda, invece, gli impegni relativamente al rapporto concessorio - quindi non sullo sviluppo della progressione societaria - le condizioni per il ripristino della piena sicurezza del rapporto fiduciario tra il concedente e il concessionario prevedono: 3,4 miliardi di euro a titolo di misure compensative; un piano di 14,5 miliardi di euro per gli investimenti sulla rete, di cui 5,5 miliardi da realizzare entro il 2024, tra l'autunno del 2020 e il 2024; il potenziamento di controlli e verifiche, e verifiche, oltre ad un aumento, e in alcuni casi al raddoppio, degli investimenti per manutenzioni sulla rete autostradale. Gli obblighi del concessionario per il riequilibrio del rapporto concessorio tra il

con un incremento massimo dell'1,75 per cento. Si prevede, inoltre, il riconoscimento del valore dell'indennizzo in caso di cessazione anticipata, come sancito da una legge del Parlamento italiano (il decreto milleproroghe del 2019, all'articolo 35), con l'applicazione del codice degli appalti e il riconoscimento dell'efficacia della risoluzione e comunque della cessazione anticipata, quando disposta, per inadempimento imputabile al concessionario con una fattispecie tipizzata. Inoltre, il pagamento dell'indennizzo in questo caso non viene

quanto prima la deliberazione del Consiglio dei ministri e addivenire alla definizione dell'accordo transattivo nei termini che ho sommariamente indicato in questi pochi minuti.

difficile immaginare il disgusto della gente a casa che sente risposte di questo tipo con le quali non si risponde in realtà a quello che si chiede. *(Applausi)*. Lei non ci ha detto quanto vale Aspi oggi, Grazie ci sarà un problema: avendo una diminuzione dei pedaggi ci sarà anche una diminuzione degli incassi, per cui non è detto che il valore di Aspi oggi sia uguale al valore di Aspi domani. Non ci ha poi detto se, agendo in questo modo, riterrà che la società sarà meno appetibile per eventuali investitori; anche questo potrebbe rappresentare un problema. Non ci ha detto chi saranno gli investitori

non pensano che sia una percezione il fatto che la Liguria e le sue autostrade siano in questo momento assolutamente isolate. Lei non ci ha detto assolutamente nulla rispetto al fatto che i giuristi da voi nominati ritenevano che le concessioni potessero essere tolte a costo zero. quindi una liquidazione piuttosto che una revoca. Avete deciso forse di confermare le tariffe invece che a rivederle. Insomma, in poche parole, ci siamo scontrati ancora con la vostra ideologia e la vostra inconcludenza. La situazione oggi in realtà - e vado a concludere, Presidente - è che chi avevate detto che doveva essere messo all'angolo oggi esce da vincitore: i Benetton infatti non escono da Aspi, ma vengono solamente ridimensionati, quantomeno inizialmente. Hanno guadagnato in questi anni godendo delle tariffe

cari compagni, alla fine siete veramente bravissimi, siete proprio di sinistra, perché state riuscendo a statalizzare le perdite e a privatizzare gli utili.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, la strategia delle tre «T» (testare, tracciare, trattare) per tenere sotto controllo il Covid-19 prevedeva anche l'utilizzo delle *app* per individuare casi positivi e isolarli. Dopo la fase di sperimentazione in alcune Regioni, la *app* Immuni è arrivata ormai da un mese su tutto il territorio nazionale. L'applicazione di *contact tracing*, già scaricabile dal 1° giugno scorso, ha il compito in effetti di tracciare gli eventuali contatti degli utenti con persone positive al al nuovo coronavirus. L'*app* Immuni permette agli utenti di telefoni cellulari che hanno attivato l'applicazione di ricevere notifica di eventuale esposizione al coronavirus. Nell'intero sistema della *app* non sono presenti, né sono registrati i nominativi o altri elementi che possano ricondurre all'identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, bensì codici alfanumerici. L'impiego dell'applicazione è volontario e operante nel pieno rispetto della *privacy* di coloro che la scaricano e ha lo scopo di aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività e di evoluzione dell'epidemia in Italia. Gli utenti di cellulari che decidono di scaricare l'applicazione contribuiscono così a tutelare se stessi e le persone che incontrano. Se sono entrati in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, vengono avvisati con una notifica dell'*app*; ciò dovrebbe consentire loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale per ricevere le indicazioni sui passi da compiere. Come risulta dai dati diffusi qualche giorno fa sugli organi di stampa, coloro che dichiarano di aver scaricato l'applicazione sono finora circa 4 milioni. di comunicazione è in corso, ma il numero di italiani che hanno scaricato l'applicazione sembra ancora essere lontano dalle soglie ipotizzate per un efficace funzionamento dell'intero sistema di tracciamento. Chiediamo pertanto a lei, signor Ministro, qual è il numero di coloro che hanno scaricato l'*app* Immuni (avrà sicuramente i dati) e quale sia il numero di soggetti contagiati. Le chiediamo soprattutto le valutazioni del Governo sull'attuale l'efficacia dell'applicazione e quali strategie di tracciamento ritenga necessario potenziare,

Signor Presidente, senatrice Boldrini, onorevoli senatrici e senatori, come è noto, dopo l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, dal 15 giugno l'*app* Immuni è funzionante in tutta Italia. L'applicazione del Ministero della salute,

Stando all'ultimo dato a me disponibile, l'*app* è stata installata da oltre 4.300.000 utenti; secondo una ricerca dell'università di Pavia, questo dato rappresenta circa il 12 per cento della popolazione italiana i settantacinque anni in possesso di *smartphone* necessari per l'utilizzo dell'applicazione. Per quanto riguarda il contributo dell'applicazione nella lotta al coronavirus, secondo il Ministero della salute i soggetti positivi in possesso dell'applicazione che hanno acconsentito all'invio del messaggio di notifica sono 46. Dal 13 luglio a oggi i soggetti allertati grazie all'applicazione risultano essere stati 23. Grazie ad "Immuni", quindi, 23 persone hanno avuto la possibilità di conoscere il rischio da contagio a cui sono state esposte. Questo dimostra l'utilità dell'applicazione. Il problema non è individuare la soglia "x" o "y" di *download* per valutare l'efficacia o meno dell'applicazione. Quando sento ripetere che l'università di Oxford ha segnato al 60 per cento la soglia minima di utilità degli strumenti di notifica di esposizione al Covid-19, mi domando perché non si legga mai il periodo successivo dello studio in questione. Permettetemi di citare, come lo riferisce la Massachusett institute of technology review: «Molti resoconti e analisi dei media hanno ripreso una frase dal rapporto, che recita: "I nostri modelli mostrano che possiamo fermare l'epidemia se circa il 60 per cento della popolazione utilizza l'*app*". Ma hanno regolarmente omesso la seconda metà della frase: "Anche con un numero inferiore di utenti dell'applicazione stimiamo comunque una riduzione dei casi di coronavirus e di decessi"». Non ho mai detto che l'applicazione sia l'unica soluzione al contenimento del virus. In Italia l'applicazione rientra in una strategia complessiva che si basa anche su altre misure di contenimento. Naturalmente più si amplierà la diffusione dell'applicazione, più sarà conosciuta e più questa sarà in grado di contribuire ad agevolare le azioni di contrasto al coronavirus. Il commissario Arcuri ha dato avvio a una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini di tutte le età circa l'utilizzo dell'applicazione, soprattutto per coloro che vivono e operano in piccoli centri urbani, all'interno delle imprese, delle associazioni, delle università e anche delle scuole. L'utilizzo dell'applicazione nelle scuole è stato suggerito dal comitato tecnico-scientifico e anche l'Ispettorato generale della sanità militare ha sensibilizzato tutto il personale delle Forze armate all'utilizzo dell'applicazione. Concludo: vogliamo che l'Italia riparta a tutti gli effetti, dai posti di lavoro, alla scuola, al turismo, vitale per il nostro Paese, e che lo faccia in sicurezza. Più siamo e più saremo a scaricare "Immuni" e più saremo in grado di spegnere nuovi potenziali focolai con vantaggi per tutti noi.

che le sue competenze rappresentino un'incidenza trasversale della digitalizzazione sull'intera nostra pubblica amministrazione rispetto a tutti gli altri Ministeri. non è quindi specifico, ma è evidente che siamo di fronte a sperimentazioni importanti, che non sono mai avvenute nel nostro Paese, che godono di accelerazioni significative in questo momento nella considerazione e nella consapevolezza dei cittadini. la soglia del successo dei *download* non corrisponde alla soglia di efficacia attesa della presenza dell'applicazione. Questo però non ci deve impedire di continuare a insistere in tale direzione e credo debba essere preso come un indice del *gap* che ancora riscontriamo riguardo non solo l'utilizzo delle tecnologie disponibili per obiettivi di servizio - c'è poi tutto un altro mondo di servizi della pubblica amministrazione che non hanno ancora incontrato i cittadini nel modo auspicato - ma anche

dal 1° gennaio al 23 luglio del 2019 ci sono stati 3.431 sbarchi; nel 2020 11.191 sbarchi. Soltanto ieri, 22 luglio, ci sono stati 689 sbarchi. Il mese di luglio 2020, fino ad oggi - non è quindi ancora terminato - registra un aumento del 223 per cento di sbarchi ed è il peggiore degli ultimi tre anni, dal 2018 alla con l'aggravante che tutto questo sta accadendo in piena emergenza sanitaria. Purtroppo i risultati nefasti della politica irresponsabile messa in atto dal Governo Conte-*bis* non hanno risparmiato la mia Basilicata. La Basilicata aveva raggiunto dopo l'emergenza Covid-19 un grande e bel primato che ci rendeva orgogliosi - essere la prima Regione Covid *free* in tutta Italia grazie al senso di responsabilità elevato dei lucani - come d'altronde di tutti quanti gli italiani - al grandissimo lavoro dei medici

Governo? Ha portato degli immigrati nei giorni scorsi, che hanno riaperto le porte dell'incubo. E questo è accaduto quando al Governo sono presenti due Ministri lucani:

da qualche giorno, 52 cittadini bengalesi, 12 in provincia di Matera e 40 a Potenza città, dei quali 10 e 27 positivi. 27 positivi. Oggi abbiamo saputo che una nigeriana, che alloggia nella stessa struttura, è positiva e fino ad ora ha girato liberamente insieme ai suoi connazionali. Concludendo, signor Presidente, il Governo deve pensare a come risarcire il danno di immagine per la Regione Basilicata: era una meta turistica sicura e l'ha ridotta - o meglio, vuole ridurla, ma non ci riuscirà - ad un lazzaretto. Non rinunceremo al sogno di una meta sicura davanti all'incapacità del Governo, così come non manderemo in fumo i sacrifici di tanti operatori turistici,

Non a caso oggi ho depositato un'interrogazione urgente al ministro Lamorgese, affinché si sappia con chiarezza perché non si sono fatti i controlli previsti allo sbarco, a Lampedusa prima e ad Agrigento dopo. Chiunque ha delle responsabilità deve essere ad esse inchiodato.

seduta è sospesa.

ore 17,07)*. Onorevoli colleghi, come già concordato in via informale tra i Gruppi parlamentari, alle ore 16,30 di martedì 28 luglio il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sulle ulteriori iniziative in relazione all'emergenza da Covid-19.